151-*bis* del Regolamento, su interventi per favorire gli investimenti a sostegno dell'innovazione e della competitività del sistema industriale italiano ed evoluzione dei negoziati internazionali sul commercio e attrazione degli investimenti esteri** che è in corso la diretta televisiva della RAI. Passiamo dunque alle interrogazioni sugli interventi per favorire gli investimenti a sostegno dell'innovazione e della competitività del sistema industriale italiano.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Ministro, il programma Industria 4.0, che il Governo ha presentato ieri, mira a ricollocare l'Italia sulla nuova frontiera delle tecnologie e a recuperare un *gap* oggi preoccupante; e consideriamo questo una gran buona notizia. Personalmente non provo particolari passioni per la distinzione filosofica tra logiche orizzontali e verticali, che pure oggi viene esaltata da «Il Sole 24 Ore». Infatti, la politica industriale le ha sempre seguite entrambe

con il CIP6 e gli incentivi alle fonti rinnovabili, che furono la più grande operazione di sussidio mai realizzata in Italia proprio mentre si diceva che la politica industriale andava bandita. Mi terrei quindi alla larga da queste e verrei invece proprio al progetto per fare un'osservazione e porle due domande. L'osservazione è che siamo davanti a un impegno finanziario di 13 miliardi spalmati su sette anni: se la politica di bilancio fosse più lungimirante, potremmo probabilmente averne di più. Le domande sono le seguenti. Posto che le tecnologie combinate dal piano Industria 4.0 sono già oggi disponibili, il loro effetto sarà nell'immediato una riduzione dei costi operativi, tra i quali spicca il costo del lavoro. Quali potranno essere, quindi, nell'immediato (nei prossimi due o tre anni) gli effetti sui livelli occupazionali all'interno delle imprese che si che si ristruttureranno e nei servizi che fioriranno loro attorno, prima che si manifestino nel medio periodo gli effetti positivi del citato piano? dalle *slide* e dalle cronache non ho capito se l'iperammortamento aumenti la base ammortizzabile dell'azienda e le aliquote reali restino costanti, o se, invece, l'iperammortamento aumenti l'aliquota reale e, dunque, riduca il periodo di ammortamento come un tempo avveniva con gli ammortamenti anticipati. In un caso o nell'altro, quali saranno gli effetti sull'utile e sulla remunerazione del capitale? Signor Presidente, signor Ministro, proprio ieri ella ha presentato Industria 4.0, un piano del Governo per un sistema industriale che innovi i propri processi produttivi e abbia accesso al mercato internazionale. Siamo in ritardo di almeno quattro anni rispetto alla Germania, dove la produzione industriale automatizzata e interconnessa è già una realtà. Ma al contempo siamo in attesa delle misure che ella ha annunciato come parte dell'articolato della nuova legge di bilancio. Mi consenta solo di ricordarle che il sistema industriale italiano industriale italiano ha però una propria tipicità: industrie di piccola dimensione, gestione familiare, prodotti di grande qualità, spesso fatti completamente a mano, appetibili all'estero, dove però è difficile arrivare da soli. È quindi certamente necessario favorire le *start-up*, dove però gli investitori hanno un orizzonte di medio periodo; agevolare le imprese che innovano, ma anche coccolare le imprese che realizzano semplicemente prodotti tradizionali, molto richiesti sui mercati internazionali. su questo tipo di imprese pesano il costo del lavoro, quello degli straordinari da pagare ai propri dipendenti quando aumentano gli ordini, ma anche quello di mantenere intatto il livello occupazionale e salariale nei momenti di crisi. allora, oltre alla annunciata riduzione dell'IRES, quali siano le misure per le aziende che non fanno utili, perché ancora non sono uscite dalla crisi, e per le aziende dove il lavoro dell'uomo è ancora un elemento predominante. inoltre, opportuno prevedere forme di incentivo fiscale all'azionariato che immette nuovo capitale nelle imprese, avendo un orizzonte di lungo periodo (almeno dieci anni), sia per le aziende quotate che per quelle non quotate? quando si parla di *patent box* pensiamo ad agevolazioni fiscali per sostenere in primo luogo la ricerca e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e la loro capacità di innovazione, premiando perciò il talento per le invenzioni e quindi i brevetti. Ma, leggendo alcuni dati diffusi dall'Agenzia delle entrate, sembra che il piano previsto dal Governo sia stato finora largamente disatteso. Il provvedimento, infatti, ha favorito più le grandi imprese e le multinazionali, creando l'ennesimo disequilibrio economico nel mercato della ricerca e dello sviluppo. Il *patent box* all'italiana, infatti, è meno restrittivo di quanto previsto dall'OCSE, che riconosce solo i brevetti come oggetto di vantaggi fiscali. Da noi, invece, si inseriscono anche i marchi, i *software* protetti da *copyright*, i disegni, i modelli e il *know-how*. I dati dell'Agenzia delle entrate parlano chiaro: delle 4.498 istanze presentate nel 2015, oltre il 55 per cento fa riferimento a società con un fatturato che va dai 10 milioni agli oltre 300 milioni di euro (tutt'altro che piccole e medie imprese, e solo il 18 per cento di queste riguardano la presentazione di brevetti. Ma non è tutto. Stando alle previsioni, il provvedimento rischia di trasformarsi in un *boomerang* per la finanza pubblica. Dei 620 milioni di euro previsti per il prossimo triennio, le quasi 4.500 domande di cui sopra ne assorbiranno circa 590 solo nel 2015, ovvero uno sconto fiscale triplo rispetto al totale dello stanziamento preventivato. Considerando, infine, che anche secondo una ricerca del Taxation and customs union della Commissione europea, nella maggioranza dei casi il nostro *patent box* ibrido produce incentivi fiscali destinati alle multinazionali senza una corrispondenza di aumento degli inventori o dell'attività di ricerca, misure intenda adottare il Governo per ripristinare una logica di equilibrio per il sostegno alla ricerca e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, nell'ottica di riportare al centro della questione la produzione dei brevetti.

Discutere di interventi a favore degli investimenti e a sostegno dell'innovazione e della competitività del sistema industriale italiano è importante, ma solo se questa discussione avviene nel quadro di una coerente politica economica, che abbia come coordinate essenziali lo sviluppo complessivo. In un contesto internazionale che mostra profondi segni di crisi e di involuzione in che modo il Governo intende affrontare questi nodi e dimostrare una coerenza che al momento non si vede? Da dove nascono queste difficoltà? Nascono soprattutto dal mutato contesto internazionale e dal ritardo con cui stiamo cogliendo l'impatto di queste trasformazioni? In estrema sintesi, signor Ministro, la crisi del 2008 con il fallimento della Lehman Brothers sembra sempre più marcare un tornante, una svolta repentina nella logica profonda che regola i processi della globalizzazione oggi in evidente difficoltà. Sarà un fenomeno temporaneo? Ce lo auguriamo. Ma le varie turbolenze non solo economiche, ma anche politiche, caratterizzate da un risorgente nazionalismo, che sconfina nell'autarchia, stanno facendo precipitare il barometro delle previsioni. E allora è necessario che l'Italia si attrezzi e rifletta sui rischi collegati a questa nuova fase si dia gli strumenti indispensabili per una diversa politica economica, all'interno della quale ricollocare gli argomenti di cui, oggi, dobbiamo discutere. Ma fino a quando non vi sarà questo ripensamento generale, rischiamo solo una discussione oziosa, che non è in grado di aggredire la ragioni più profonde della crisi italiana. Signor Presidente, ieri è stato presentato Industria 4.0, il piano per rilanciare il nostro sistema industriale con una serie di misure per promuovere investimenti e innovazione. Incentivi fiscali, rafforzamento degli strumenti finanziari e collaborazioni con le università: sono esempi di misure sicuramente opportune e degne di apprezzamento. Apprezziamo che il Ministro abbia più volte sottolineato la necessità di intervenire in questo campo. È indispensabile, però, ricordarsi di agire con aumenti importanti degli investimenti pubblici e privati. Lo diciamo pensando che il Paese è ancora in dietro su molti aspetti che non possono privarsi di tali strategie. Ad ogni modo, pensiamo che il piano presentato ieri sia più che altro un bel libro dei desideri. Troppi sono i riferimenti a modelli di sviluppo decisamente lontani e inapplicabili. Troppo è il peso che si affida al concetto di flessibilità. È chiaro - e lo sappiamo tutti - che bisogna sviluppare l'innovazione e farlo guardando al futuro. Quel piano, però, non sembra tener conto delle caratteristiche strutturali del Paese. Mi riferisco in particolare alla struttura organizzativa delle imprese e del sistema socioeconomico italiano. Penso al settore dei servizi e ai limiti ancora causati dalla scarsa apertura al mercato. Penso al *caos* di leggi e regolamenti che carica ancora di enormi costi chi fa impresa. Penso ai tempi lenti della burocrazia. E soprattutto, cari colleghi, penso che la somma di tutte queste autentiche ferite sia ciò che ancora oggi fa scappare le grande aziende straniere dal bel Paese. Chissà quante opportunità e quanti posti di lavoro avremmo se superassimo una buona volta questi ostacoli. Ci vuole, però, una volontà politica che qui non trovo. Il presente piano, quindi, anche se parte da buone intenzioni, non va a curare le cause reali dei problemi e probabilmente separa ancor di più il Nord dal Sud. In conclusione, Presidente, da parte nostra esistono diverse zone d'ombra e molte domande che chiedono urgenti risposte, a iniziare dalle risorse, fino alla scelta delle modalità di attuazione. Quali sono i provvedimenti che agiscono su costo del lavoro e riduzione fiscale? Perché non si insiste realmente sullo sblocco dell'Alta velocità anche nel Mezzogiorno?

economico*. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli argomenti sono ovviamente molto interconnessi e per questo mi permetto di rispondere congiuntamente per poi andare nello specifico.

più cause non sempre collegate che si mettono insieme (prezzo delle materie prime, svalutazioni, instabilità geopolitica). In questo contesto,

non tutto va bene per gli investimenti pubblici e non tutto va bene per gli investimenti privati. Il piano che abbiamo presentato ieri lavora sullo stimolo soprattutto agli investimenti privati.

Vengo alle cose specifiche. Non sono appassionato neanche io al dibattito tra orizzontale e non, ma il tema sollevato da molti di voi è relativo all'accesso delle piccole e medie imprese. È del È del tutto evidente che incentivi fiscali automatici funzionano molto meglio per una piccola e media impresa rispetto a un incentivo - per esempio - a bando, che diventa complesso e ha tempi di attraversamento molto lunghi. I 13 miliardi non sono per sette anni, perché perché in tutta la parte di iperammortamento e superammortamento coprono gli investimenti effettuati nel 2017. Questo vuol dire che, anche dal punto di vista puramente di uso delle risorse pubbliche, si ha un'anticipazione degli effetti e un esborso nel tempo.

privi dei posti di lavoro. L'altro elemento è l'aumento della produttività, che fa sì che la variabile del costo del lavoro - è una delle variabili che ha spinto alla delocalizzazione - diventi meno influente. Queste sono due cose che potrebbero equilibrarsi. Con il ministro Poletti ieri

Allo stesso modo stiamo lavorando - è una questione che attraversa i vari interventi - su un potenziamento ulteriore dell'incentivo al salario della produttività. Il pezzo di salario collegato alla produttività è quello che, sempre di più, con questo tipo

Molto spesso la domanda interna è una fiammata che si spegne rapidamente e non costituisce la premessa per avere anni di crescita. Tra gli altri strumenti che stiamo utilizzando c'è una forte riforma dei contratti di sviluppo. Ricordo che l'80 per cento va al Sud. Ci abbiamo messo sopra un miliardo di euro.

fatto riferimento a misure che erano state prese e che l'Unione europea - per esempio - ha invalidato. Abbiamo avuto di recente una *comfort letter* della Commissione che approva il nuovo schema sugli energivori, che promulgheremo il prima possibile.

per cento delle domande proviene da imprese che hanno meno di 10 milioni di euro e io penso che questo sia un risultato molto importante. Non dobbiamo ragionare sugli elementi della crescita nel senso che uno sia da privilegiare rispetto a un altro; stanno insieme. Se noi attraiamo investimento ad alto livello di ricerca e innovazione delle multinazionali, non è un fatto negativo, ma positivo, visto che intorno vivono ecosistemi di piccole imprese. Se le aziende medie, quelle cioè attorno ai 10 milioni di euro, incominciano a lavorare di più sulla frontiera dell'innovazione - e questo è anche il piano Industria 4.0 - è un fatto positivo anche per quelle molto più piccole, che spesso proprio da fornitori diventano poi più grandi. Credo che dobbiamo dunque ragionare su una platea di imprese e su una platea di strumenti, ciascuno dei quali abbia un suo *target*. Il piano Industria 4.0 è fatto per le piccole e medie imprese perché ha quell'automatismo che a loro serve, anche nel credito d'imposta per ricerca e innovazione, che abbiamo potenziato

che reputo molto importante: mi riferisco al fatto che la società che sponsorizza e investe in una *start-up* possa prendere le perdite della *start-up* e portarsele sopra. Quello che oggi sta succedendo nel mondo è che spesso la ricerca e l'innovazione non vengono più fatte solo internamente, ma anche attraverso la partecipazione di *start-up.*

può rispondere a tutte le esigenze che il Paese ha in termini di crescita? Ovviamente no. Non è costruito per questo. Non è costruito per essere onnicomprensivo. È costruito per lavorare sui fattori di competitività dell'impresa. Poi, certo, ci vogliono l'alta velocità, gli investimenti pubblici, e ne stiamo facendo alcuni molto qualificanti - penso a quello della banda larga - ma questo è il è il pezzo che ci assicura una crescita duratura. Il punto è riuscire a portare le aziende con strumenti facili, concentrati e di una magnitudine sufficiente dentro questa rivoluzione. Noi siamo anche grandi produttori di macchine utensili: esportiamo più macchine utensili e automazione di tutti gli altri principali settori del *made in Italy* messi insieme. Per tale motivo questa rivoluzione è un rischio, ma anche una straordinaria opportunità. Se noi riusciremo ad agganciare questa manovra al filone di innovazione e competitività del sistema imprenditoriale italiano, quel pezzo sarà fatto. Come ultimo punto di filosofia, abbiamo dato degli strumenti alle imprese. Sta alle imprese adesso utilizzarli. Non sono strumenti per cui devono chiedere a nessuno un timbro: devono fare, investire. Questo è quanto devono fare loro. Certo, tutto questo presuppone una fiducia nel mondo imprenditoriale italiano e da parte del Certo, questo presuppone il fatto che il mondo editoriale italiano abbia la spinta ad innovare, ma non credo che ci sia una strada differente da quella che stiamo imboccando, sapendo che i prossimi anni rimangono di grandissima incertezza e, come tali, vanno attraversati. Ma non c'è una strategia diversa da questa; anzi, più incertezza c'è, maggiore è lo stimolo agli investimenti, che sono l'unica risposta vera all'incertezza che noi dobbiamo dare.

ringrazio per la risposta, della quale prendo atto, e mi riservo nel prosieguo - anche in occasione della sua audizione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato - un ulteriore approfondimento del tema.

innovazione tecnologica e digitale. Sul premio alla produttività bisognerà verificare se le risorse annunciate ci saranno. Ci sembra, però, veramente minimo l'intervento a sostegno del *made in Italy*, tra l'altro in un momento in cui esso subisce ogni tipo di attacco da parte di prodotti fatti all'estero e spacciati per italiani. Ci pare che al suo Governo manchi ancora una visione ampia sul mercato dei capitali, ed è assente anche un serio piano per il sistema creditizio all'economia reale. Mi auguro, quindi, che voglia accogliere

Bastava ammettere semplicemente che, come fa il resto dei Paesi OCSE, non andavano inseriti i marchi e gli altri oggetti che non fanno veramente ricerca e innovazione. È il brevetto fa ricerca, innovazione e sviluppo, e non i marchi, che è tutta un'altra cosa: è solo *marketing*. Comunque sia, ribadisco la conclusione - non mia o del Movimento 5 Stelle, ma della Commissione europea secondo cui questo tipo di regime, *patent box* italiano, ha spostato semplicemente la sede delle multinazionali che, per approfittare dello sconto fiscale, vengono registrate in Italia. Quindi, quel 44 per cento a cui faceva riferimento lei non è comunque frutto di attività locali,

*(AL-A)*. Signor Ministro, è lei che ha parlato di filosofie, quindi, mi ha autorizzato a fare un esempio: quello del papà di famiglia che ha radunato attorno al tavolo tutti i suoi figli e gli ha spiegato la filosofia, la cultura e la politica, la politica, e il più piccolo, all'ultimo, condividendo l'intervento del padre, gli ha chiesto: «Ma questa sera che cosa mangiamo?». Signor Ministro, riusciamo a capire le sue difficoltà: il Dicastero non può stare con le mani in mano in attesa che dal Consiglio dei ministri giungano le risposte necessarie ai temi che ha sollevato. a capire un certo imbarazzo, ma la consapevolezza delle difficoltà che ci attendono dovrebbe spiegarci e farci promotori delle necessarie iniziative e, quindi, creare effettivamente i presupposti affinché gli investimenti a sostegno dell'innovazione e della competitività del sistema industriale italiano si realizzino Il Governo sprona gli industriali, ma gli industriali non si fidano di questo Governo e del sistema che li sta circondando, ivi compresi i problemi giudiziari che investono tutti gli investitori italiani, che hanno veramente paura.

che si possano sanare i punti poco chiari e che l'innovazione - per il bene di tutti - non sia solo una bella parola per rendere interessanti i programmi nell'agenda del Governo.

Signor Ministro, il Governo italiano ha più volte espresso una posizione favorevole alla conclusione del negoziato sul Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, che prevede la creazione di un'unica area di libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti. Dalle valutazioni sull'impatto economico del TTIP - con particolare riferimento a quelle prodotte dalla Commissione europea - si evince che il Trattato può rappresentare un importante volano di crescita per per l'economia europea e italiana. Tuttavia, da più parti sono emerse preoccupazioni per i potenziali impatti negativi su alcuni settori nonché sui diritti dei lavoratori e sul diritto degli Stati a regolamentare. Il Governo italiano ha più volte ribadito che il Trattato in questione può, al contrario, essere un'occasione per garantire adeguata tutela ai prodotti italiani sui mercati internazionali e prevenire forme di concorrenza sleale. Domando al Ministro in quale modo il trattato potrà favorire l'economia italiana, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e quali sia lo stato dell'arte della negoziazione. ha facoltà. PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, l'attrazione degli investimenti esteri in Italia riguarda, in modo prioritario, le aziende italiane che, di norma, abbiano un *target* internazionale per i propri prodotti. Gli investimenti esteri in Italia negli ultimi anni sono stati orientati soprattutto sulla partecipazione in grandi imprese o banche di grandi dimensioni a prezzi di saldo. Diverse operazioni sono state, infatti, portate avanti approfittando della crisi economica e del conseguente crollo La cosa positiva è che si tratta, in alcuni casi, di investitori di lungo periodo; la cosa negativa è che si è comunque «bruciato» capitale italiano. Non è stata, quindi, aggiunta alcuna ricchezza. Purtroppo, quello che va sottolineato è la presenza di un saldo negativo tra investimenti italiani all'estero e investimenti esteri in esteri in Italia; così come è comunque negativo quello degli investimenti di portafoglio. Sono sempre di più i capitali italiani che vanno all'estero rispetto a quelli esteri che vengono investiti in Italia. Si aggiungano a questo i denari e il *know-how* di imprese italiane che delocalizzano le proprie produzioni portandole all'estero. Il risultato è quindi un prodotto interno lordo che cresce meno delle aspettative. Signor Ministro, le chiedo allora: ancor prima di attirare investimenti dall'estero non ritiene che sarebbe più saggio fermare i capitali, gli imprenditori e le imprese italiane che vanno all'estero? In questo senso, l'azione solitaria del suo Ministero non è sufficiente, ma serve quel quadro di regole da sempre evocato: meno burocrazia, più credito, giustizia più veloce, meno tasse. *(M5S)*. Signor Ministro, i negoziati su trattati come il CETA o il TTIP si sono svolti nella più assoluta segretezza; non è stato possibile un reale controllo da parte dei rappresentanti democraticamente eletti né un confronto con la società civile. Ricordo a tutti che questi trattati riguardano l'assetto commerciale e produttivo e sono trattati in cui l'Italia, secondo molti, ha tutto da perdere. Addirittura, il CETA potrebbe entrare in vigore con un trucco, quello dell'applicazione provvisoria, ossia senza che i Parlamenti nazionali ed europeo possano ratificarlo o respingerlo. Pertanto, signor Ministro, sono a chiederle se il Governo italiano vuole favorire l'approvazione nei vari Parlamenti nazionali di un trattato come il CETA oppure avalla questo trucco dell'applicazione provvisoria. Sul TTIP, invece, visto che Francia e Germania ed altri Paesi europei che in totale fanno una rappresentanza di oltre il 56 per cento della popolazione europea vanno verso uno stop alle trattative, chiedo perché l'Italia vuole invece forzare la mano - almeno pare - su un tavolo da cui, ripeto, molti ci dicono che ha tutto da perdere.

lei rispondeva, senza esitazioni, che il negoziato sarebbe proseguito e ribadiva la posizione del Governo favorevole al raggiungimento dell'accordo, affermando che cito testualmente - questo è il modo per riprendere in mano il timone della globalizzazione. Il nostro Parlamento e quelli di altri Paesi membri hanno già espresso, a più riprese, proteste formali per la scarsa trasparenza con la quale sono state condotte le trattative e per la mancata e tempestiva circolazione dei documenti, a partire dagli aspetti più controversi oggetto di confronto nei diversi tavoli negoziali. Ne cito solo alcuni: dalle norme europee su OGM, etichettatura e pesticidi, agli *standard* previsti nei settori energetici, alla chimica. Penso all'assenza negli Stati Uniti del principio di precauzione per cui, per esempio, le sostanze chimiche sono considerate sicure fino a prova contraria; penso alla riduzione in generale degli *standard* sociali ed ambientali. A fronte dell'esplicita richiesta di sospensione formulata dal Governo francese e dell'altrettanto esplicita ammissione di fallimento proveniente dal Ministro dell'economia tedesco, ci sembra indispensabile che il Parlamento e l'opinione pubblica ricevano oggi una chiara informativa sulla posizione ufficiale del Governo italiano al tavolo negoziale sullo stato reale delle trattative. È a lei senz'altro noto che ci sono settori dell'economia nazionale che verrebbero pesantemente investiti dalle conseguenze di un eventuale accordo sul TTIP. Mi riferisco, in particolare, al comparto agroalimentare e non solo. Voglio inoltre chiederle se, ad oggi, è stato adeguatamente valutato l'impatto occupazionale che un eventuale accordo avrebbe sull'economia del nostro Paese. Mi riferisco, in particolare, al documento pubblicato dalla direzione generale per le politiche interne del Parlamento europeo quattro mesi fa, in base al quale il nostro Paese, insieme alla Germania, sarebbe il più colpito dalle conseguenze del TTIP, con una stima di 300.000 posti di lavoro a rischio. Analoghe assicurazioni le chiedo in merito all'accordo di

dei negoziati internazionale sul commercio tra le due sponde dell'Atlantico non è altro che una conseguenza della nuova fase che sta caratterizzando il processo di globalizzazione, il cui rallentamento non può che preoccupare, non essendo ancora disponibile un piano B per far fronte ai più limitati impulsi del commercio internazionale. Ben diverso è, invece, il caso delle politiche rivolte all'attrazione degli investimenti esteri, dove alcune patologie stanno determinando allarme nell'opinione pubblica, non solo italiana. Mi riferisco, in particolare, alla vicenda della Apple e dei suoi privilegi fiscali in terra d'Irlanda, che hanno costretto la Commissione europea ad intervenire duramente. Ricordo che prima c'erano stati il caso della Volkswagen e la multa miliardaria decretata dagli Stati Uniti. C'è un caso meno noto su cui vorrei richiamare la sua attenzione, signor Ministro. Si tratta di un caso ancora più scandaloso dal punto di vista etico, perché riguarda la vita di due milioni di malati, quelli colpiti in Italia dall'epatite C. L'epatite

Il ciclo completo ci costa 40.000 euro, cifra insostenibile sia per il singolo, sia per il Sistema sanitario nazionale. La cosa che fa discutere è che lo stesso farmaco ha un costo di 800 euro

dovuto godere di una cura *gratis*. Signor Ministro, le segnalo il caso, non tanto per i risvolti sanitari, di cui discuteremo in altra sede, ma per quelli più propriamente economici e finanziari. Sul banco degli imputati non ci sono solo la Volkswagen e la Apple. È infatti evidente che fin quando un fronte comune rispetto alle politiche praticate dalle multinazionali, con regole certe e uniformi nell'attrarre investimenti, saranno i Paesi più egoisti ad avere la meglio. LIUZZI *(CoR)*. Signor Ministro, secondo le valutazioni più recenti, peraltro ricorrenti in questo dibattito, il nostro Paese, su una scala di attrattività per un investitore straniero,

investimenti la nostra economia langue. Ma che cosa scoraggia davvero gli investitori internazionali? Quasi a voler suggerire una risposta a questa domanda, il Governo incoraggia l'approvazione in tempi brevi dei due accordi economici e commerciali fra l'Unione europea e il Canada (CETA) e quello fra l'Unione europea e gli Stati Uniti (TTIP). Il CETA ha concluso la fase negoziale e, se venisse approvato entro la fine del 2016 da Consiglio e Parlamento europei, potrebbe entrare in vigore nel 2017. Lei, signor Ministro, addirittura auspica la ratifica direttamente da parte del Parlamento europeo senza la previa approvazione dei singoli Parlamenti degli Stati membri. Indipendentemente dal fatto che ciò sia giuridicamente corretto (ma ci sembra che non lo sia), nel frattempo i cittadini di tutta Europa si riuniscono per manifestare contro l'approvazione di questi questi trattati dai molti lati oscuri, tra i quali il timore che si voglia favorire, volenti o nolenti, tanto con il CETA, quanto con il TTIP, gli interessi delle multinazionali a scapito di quelli dei cittadini. È inoltre opinione diffusa che, dai negoziati ormai conclusesi per il CETA si poteva ottenere molto di più, soprattutto in termini di maggiori garanzie per la salute dei consumatori europei. Non a caso Paesi come la Germania e l'Austria non daranno via libera al CETA senza che sia stato prima approvato dal Parlamento nazionale. Ma al di là di questo tipo di rivoluzionari accordi internazionali, l'inadeguatezza del nostro Paese sul piano dell'attrattività per i nuovi investimenti viene da lontano e riguarda il funzionamento della macchina pubblica. Sono la pubblica amministrazione e le sue inefficienze a preoccupare maggiormente gli investitori. Le chiediamo, perciò, signor Ministro, quali misure stia predisponendo il Governo per aumentare la puntuale conoscenza dei contenuti dei due Trattati da parte dei cittadini e in particolar modo delle imprese italiane al fine di garantire la tutela dei nostri marchi e delle nostre produzioni tipiche e di eccellenza e, nel contempo, quali misure si intendano

il rapporto tra le nostre esportazioni e il PIL è del 30 per cento a fronte di quasi il 50 della Germania.

mentre invece molti altri Paesi, Stati Uniti compresi, lo sono molto meno. Dunque rimanere fermi, per l'Europa, non è la soluzione. Aggiungo questo: gli Stati Uniti oggi sono uno dei nostri mercati più importanti, il terzo in assoluto, con una crescita molto significativa: esportiamo 36 miliardi di beni ma soprattutto facciamo 22 miliardi di euro di saldo positivo.

Ora, su questo è girata una informazione molto scorretta e visto che, giustamente, ci lamentiamo del fatto che ci vuole più trasparenza sul Trattato, vorrei dire che, in qualità di presidente del consiglio del commercio ho desecretato, per la prima volta nella storia dei trattati commerciali, il mandato negoziale sul TTIP. TTIP. In questo mandato, obbligatorio e dato all'unanimità, è chiarito che non muta il principio di precauzione, non si può negoziare, cioè, il principio di precauzione che è la base giuridica su cui noi teniamo fuori la maggior parte degli OGM. Non solo: dopo l'inizio dei negoziati abbiamo emanato anche una regolamentazione che consente anche agli Stati nazionali di regolamentare.

affinché riconoscano le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Dunque, parliamo di questo Trattato (e non è detto che lo vogliamo concludere: lo concluderemo solo se le condizioni saranno positive per l'Italia), ma facciamolo in termini corretti e non in termini che nulla hanno a che fare con il negoziato in corso. È vero che questo negoziato non ha avuto sufficiente trasparenza, ma è anche vero che nessun negoziato prima di questo ha avuto tale grado di trasparenza. Per nessun negoziato è stato consentito di visionare testi non ancora stabilizzati, che sono solo proposte negoziali: al Ministero abbiamo aperto una sala, davvero poco frequentata - se posso dirlo -, per consultarli.

scarse le possibilità che si chiuda nell'Amministrazione Obama, ma ciò non vuol dire revocare il mandato alla Commissione. È un altro discorso: vuol dire vedere se c'è l'opportunità politica. Certo, senza un riconoscimento

più di uno in molti Paesi. Ciò mi porta a parlare del CETA, che è un accordo di natura completamente differente. Del CETA abbiamo il testo e sappiamo cosa contiene: intanto c'è un riconoscimento, per la prima volta in un Paese anglosassone, delle indicazioni geografiche. Il prosciutto di Parma entrava in Canada come «*original* prosciutto», adesso può entrare come prosciutto di Parma e questo vale per tantissime altre categorie. Inoltre abbiamo un accesso al *procurement* che gli Stati Uniti non ci danno, invece in quel caso

La Commissione, sotto la spinta degli Stati membri, ha deciso di portarlo come accordo misto, quindi soggetto a ratifica nazionale, in quel processo che abbiamo descritto prima: si tratta di un processo pericoloso, perché non se ne conoscono gli esiti. Al momento è ancora giuridicamente poco chiaro cosa succede se un singolo Paese non ratifica l'accordo. L'applicazione provvisoria vale per tutta la componente del Trattato che è sicuramente *EU only* ed è stata fatta in tutti gli altri accordi.

se non negoziamo con una massa critica e soprattutto se le nostre controparti sanno che quando negoziamo poi il Parlamento vallone potrebbe bocciare l'accordo per tutti quanti. Questa è una domanda che dobbiamo farci. Il Governo italiano su questo ha preso una posizione molto europeista e non possiamo essere europeisti a giorni alterni, cioè dirlo in teoria e poi non esserlo non esserlo in pratica. Il tema dell'attrazione degli investimenti nelle vostre domande assume contorni molto differenti. Non vogliamo far venire le multinazionali, ma vogliamo attrarre più investimenti: delle due l'una.

ed è inevitabile che lo facciano. Mi stupisco che venga da lei la richiesta di limitare la circolazione dei capitali (tra l'altro, è contraria a qualunque norma europea e difficilmente praticabile). Dunque dobbiamo scegliere qual è la nostra linea. La linea del Governo è che ciò che importa non è la proprietà, ma il luogo dove l'azienda sta, dove dà lavoro, dove fa ricerca e innovazione; certe volte questi elementi sono anche rilevanti, ma il principale è sapere e su questo ci muoviamo. Per attrarre investimenti non esistono politiche diverse da quelle di cui abbiamo parlato, quelle di contesto, di produttività totale dei fattori, di costo dell'energia, di riforma della giustizia; non c'è una strategia che può accelerare tale processo. Siamo un Paese relativamente poco attraente, perché negli anni abbiamo trascurato di essere un Paese facile per le industrie. Cambiare questo percorso è l'impegno del Governo; è questo il modo in cui si attraggono gli investimenti, mantenendo in noi

Signor Ministro, mi dichiaro soddisfatta, ma auspico che anche nel prosieguo delle trattative si tenga conto dell'esigenza di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, tanto nelle esportazioni fuori dall'Unione europea, quanto sul versante interno, garantendo i consumatori sull'origine e la qualità dei prodotti commercializzati in Italia. Anche nella mia qualità di componente della Commissione agricoltura e di relatrice, nella Commissione medesima, sull'affare assegnato n. 440 in materia di strategia commerciale dell'Unione europea, ritengo infatti che il *made in Italy* debba essere supportato e protetto a tutto campo, in particolare il comparto del *food*, che registra già ora un andamento soddisfacente. *(FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, purtroppo il dato degli ultimi tre anni (che coincidono con quelli del Governo Renzi) mostra un aumento di circa 150 miliardi di euro degli investimenti italiani all'estero e una diminuzione di 28 miliardi degli investimenti esteri in Italia. Ribadiamo quindi che non è solo un problema di politica industriale, ma anche di politica economica e di saper governare a casa nostra la politica monetaria che, come lei sa bene, viene decisa a livello europeo. Ci attendiamo da questo Governo un'azione molto più forte e incisiva su tutto il comparto industriale, tale da riportare il nostro Paese tra i più grandi competitori internazionali.

Questo si potrebbe tradurre in un condizionamento delle leggi dell'Unione europea a opera di imprese e Governi stranieri prima ancora che rappresentanti europei eletti ne giungano a conoscenza. Le assicuro che si possono fermare sia il CETA che il TTIP ed è già dimostrato. In Germania hanno già cominciato a parlare di morte del TTIP, mentre il Presidente francese sta perfino chiedendo una fine formale delle trattative. Naturalmente, nella logica dell'ipocrisia, allo stesso tempo accelerano ulteriormente sull'accordo con il Canada perché tutti, *lobby* delle imprese dietro di loro, possano ottenere attraverso il CETA quasi tutto ciò che si aspettavano dal TTIP. Pretendiamo che si prenda una posizione chiara e decisa sui punti critici, senza cantare inni privi di senso sui benefici del commercio. E visto che ho ancora qualche secondo, mi spiace che lei ad esempio non abbia toccato l'inversione dell'onere della prova. Toccherà al cliente dimostrare la nocività eventuale di un prodotto contro una grande multinazionale, forse. Chissà come va a finire. [DE Signor Presidente, certamente non posso ritenermi soddisfatta. Lei, Ministro, è venuto qui a magnificare gli effetti positivi del TTIP,

quello che accadrà sia per quanto riguarda il Consiglio per la cooperazione regolativa, che è l'organismo che ancora oggi nei trattati è chiamato a fissare gli *standard* transatlantici di libero scambio, quindi scavalcando i Parlamenti, sia per quanto concerne l'organo di arbitrato internazionale, costituito da arbitri scelti con metodi extragiudiziali, che sarà chiamato a decidere sulle controversie tra investitori privati e i Paesi aderenti. Le multinazionali potrebbero cioè accusare gli Stati di intralciare il libero mercato. Questi sono i punti, perché a parole i benefici si possono decantare e anche l'ipotetico aumento dello 0,5 del PIL, ma sui dati invece bisogna essere precisi, così come su questi elementi giuridici che sono molto oscuri e saranno molto svantaggiosi per il nostro Paese.

Lei si renderà conto che il nostro Gruppo le vuol mettere a disposizione 60 miliardi per lo sviluppo economico. Da dove prenderli? Da questo accordo segretato tra AIFA e la multinazionale americana che ha fissato il prezzo a 38.000 euro. La stessa società farmaceutica con l'Egitto, con il Ministero della salute, lo fissa a 800 euro. Lei risparmia 60 miliardi. Capisco il suo imbarazzo, ma il farmaco è lo stesso. Fa guarire ugualmente. Signor Ministro, non possiamo avere uno Stato che fa la faccia feroce contro i farmacisti o i tassisti nella giusta difesa dei principi della concorrenza e della liberalizzazione e poi si volta dall'altra parte quando dall'altro lato del tavolo ci sono multinazionali che speculano sulla salute degli ammalati. può esistere in una Repubblica democratica. È per questo che noi le mettiamo a disposizione i 60 miliardi di sua competenza per cercare di

ha ragione quando parla di complessità dei contesti negoziali del TTIP e del CETA, specialmente quando si riferisce alla questione degli *standard*. Ma mi consenta di suggerirle, a proposito del fugare il campo dai sospetti, particolare sulla funzione delle multinazionali, di aumentare il livello di informazione sugli operatori economici, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni datoriali e ovviamente delle Camere di commercio a livello provinciale, al di là della stanza dei bottoni allestita presso il Ministero. Probabilmente questa azione più coinvolgente e capillare potrebbe servire allo scopo. Come pure per aumentare il grado di appetibilità delle imprese italiane, lei autorevolmente, dall'interno del Governo, può sicuramente incidere su azioni virtuose, in primo abbreviare i tempi della giustizia civile, in secondo luogo per abbreviare i tempi di riscossione dei crediti da parte delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e, infine, per poter dare, appunto, alle imprese tempi certi in tutti i sensi.